in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

alla luce di quanto emerso negli ultimi tre giorni sui giornali, dove si sono espressi autorevolissimi e qualificati esponenti del mondo ebraico

non mi sembra che questo tipo d'impostazione abbia raccolto molte adesioni, anzi, direi che ha raccolto la sostanziale unanimità dei dissensi, che si sono divisi tra quanti non chiedono nessun tipo di norma

scritto in maniera più adeguata agli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Signor Presidente, a differenza di chi mi ha preceduto, non mi sento di dare troppa importanza

del Presidente della Commissione, neanche formalmente del relatore o del Governo, che riscriveva completamente il dettato normativo. Su questo è stato condotto, direbbe il collega Zanda, un mini ostruzionismo da parte di qualche senatore dell'opposizione. Vorrei chiedere soltanto la sua valutazione, a prescindere dal merito del provvedimento cui si richiamava il collega Giovanardi,

completamente la legge, l'opposizione abbia non già il diritto ma direi il dovere di appellarsi alla Presidenza e allo stesso Presidente della Commissione per valutare

tutti - non furono molti: sei o sette - svolti nella seduta di martedì pomeriggio elogiavano il lavoro in Commissione che aveva portato a quel testo e, come vede, prescindo dalla sgradevole e sguaiata intervista di un esponente della Camera che accusava i senatori in Commissione di avere stravolto la legge. Ne prescindo perché quando il Senato delibera sarebbe elegante che da parte della Commissione giustizia della Camera vi fosse l'identico rispetto che c'è da parte nostra quando in

questo mi sembra un emendamento fondamentale. Non a caso, chi fuori dal Senato sa leggere e scrivere

il termine «diffusione» non era preciso, passò il termine «propaganda»; anche la senatrice Finocchiaro Fidelbo lo ricorderà, perché intervenne in quel dibattito. il termine «propaganda».

dell'idea che viene testimoniata. Se permettete, chi è intervenuto ha scritto: «Ma che cosa state scrivendo?». Stiamo facendo delle leggi, non stiamo scherzando. Si è inoltre scoperto - salvo che qualcuno autorevolmente lo smentisca - che con questa norma puniremo migliaia di casi di negazionismo.

e anche di coloro che sono rimasti dall'altra parte di quello che una volta era il confine dell'ex Jugoslavia. Quante volte con loro ci siamo appassionati e ci siamo anche cimentati, di fronte a una storiografia

in riferimento ai settori più oltranzisti di quel mondo, che la storiografia slovena o croata che nega le foibe non la si combatte denunciando e mandando in galera la Kersevan, che ha tutto il diritto di scrivere la sua interpretazione storica di quel periodo e che va confutata con dei dati certi. sempre per approfondire queste tematiche, sono andato a vedere il comportamento degli italiani in Slovenia nei due anni in cui venne annessa la provincia di Lubiana, mi è sembrata esagerata

come è una verità storica quella delle foibe, quella terribile pulizia etnica o ideologica che è stata fatta al di là del confine. Ma sono il dibattito storiografico e la coscienza dei giovani ciò che emerge dalla conoscenza di questi fatti, che devono rintuzzare questo negazionismo. In questo disegno di legge condanniamo a pene severissime chi nega questi fatti ma non chi li esalta; non c'è l'aggravante per l'esaltazione.

a compiere determinati misfatti, crimini di guerra o genocidi, non ho l'aggravante. Qualcuno mi faccia il piacere di spiegarmi come si farà il 10 maggio, quando tutti gli storici italiani si troveranno a Milano a discutere di negazionismo: lì ci sarà il fior fiore della storiografia italiana che si confronterà con le cose che abbiamo scritto in

cosa serve chiamare la società civile, gli storici, gli intellettuali, sentire la loro opinione e poi fare esattamente il contrario di quello che ci chiedono, dicendo che così li tuteliamo? Ma come li tuteliamo? Così li danneggiamo, annacquando l'Olocausto in altre migliaia di fattispecie che con esso non hanno nulla a che fare! L'Olocausto è l'unica volta nella storia dell'umanità in cui su scala industriale si è tentato l'annientamento di un intero popolo. E se la guerra non fosse finita come è finita, quel disegno probabilmente si sarebbe compiuto; qualcuno, ancora oggi, mentre parlo, lo vuole compiere. Vi ho letto l'altro giorno le dichiarazioni di Stati sovrani

l'esaltazione di questi fatti. Il fatto poi che ciò non modifichi il giudizio negativo su tutta l'intelaiatura del provvedimento è sicuro, ma almeno non incorreremmo in

Forza

lasciando intatto il resto dell'emendamento, che verrebbe a costituire l'intero disegno di legge, limita

Conosciamo l'*iter* travagliato di questo provvedimento: approvato in un modo al Senato, poi radicalmente cambiato dalla Camera, nuovamente modificato in Commissione e, ancora una volta, cambiato - ora - in Aula con un emendamento. ne ha cambiato molto la fisionomia sia rispetto a quanto approvato dalla Commissione pochi giorni fa, sia rispetto a quanto aveva approvato il Senato in sede di prima lettura. Mi piacerebbe sapere, ma temo che questa richiesta resti sospesa nel nulla, perché si ritiene di esprimere parere contrario a questo emendamento, e quali sono gli altri fatti storici che s'intende opportuno inserire in questo provvedimento, che ha tutta la delicatezza di essere sul filo - a mio parere

chiamiamola così, ma in questo caso è una mostruosità - viene usata nell'ambito dell'incitamento all'odio o alla violenza. Mi piacerebbe però sapere quali sono gli altri episodi che si vogliono includere,

diritto di saperlo, visto che ci troviamo, se non fosse per i subemendamenti, con un solo voto a decidere dell'intero provvedimento. per sostenere l'opportunità di introdurre questa aggravante della negazione della Shoah vale - e mi pare che lo si è sempre detto - per l'aspetto specialissimo che ha questo orribile fatto storico. Altri fatti, altri crimini di guerra, inclusi nell'amplissima definizione degli articoli 6, 7 e 8 del trattato con cui si istituisce il Tribunale internazionale e non rispondono a questi criteri, e lì davvero rischiamo di andare non verso un reato di opinione, ma verso una ingessatura, una stigmatizzazione dell'approfondimento storico su tantissimi fatti che possono andare fino ad episodi del tutto marginali dal punto di vista storico. Intendiamoci, un crimine di guerra è sempre una cosa orribile, ma una sanzione di questo genere era giustificata dal fatto unico ed eccezionale, nella sua brutalità e nel orrore, come lo sterminio degli ebrei da parte del regime nazista e di regimi suoi alleati, che è quello al quale il mio emendamento riporterebbe l'oggetto dell'intero disegno di legge. Mi sembra opportuno, se non altro per capire il perché: si può anche votare contro il mio emendamento per un buon motivo, ma sarebbe interessante sapere qual è.

come e quanto lui, ascolterei con molto rispetto da parte della Commissione e del Governo le ragioni che hanno portato a non accettare quel punto di vista tanto storiografico quanto del senso comune. Quale punto di vista? L'unicità e l'irripetibilità della tragedia della Shoah. Se da parte di qualche collega si dice «Sì, in passato si è pensato così,

allora credo che il Parlamento abbia tutto il diritto di sapere perché. Respingere in silenzio senza motivazioni l'emendamento del

dell'esaltazione della Shoah, del diritto a distruggere il piccolo satana, lo Stato d'Israele, il proprio biglietto da visita. Il nostro Governo si è recato in visita; ha guidato un'ampia delegazione di Confindustria ed ENI. *Les affaires sont les affaires*, e non solo. Proprio per questo sarebbe stato perlomeno decente che, venti giorni dopo, a un'opposizione che non aveva fatto alcun atto di sciacallaggio si dicesse perché

e, nel momento in cui si parla di negazionismo, annacqua quella cosa, unica nella storia dell'umanità, facendola confondere con migliaia e migliaia di casi.

questi argomenti - dico che mi fa molta impressione sapere che chi vota questa legge mette esattamente sullo stesso piano lo sterminio di 6 milioni di persone

troverete che il crimine di guerra, di cui si nega l'esistenza sulla base di un concetto di superiorità - quello che gli arabi addebitano agli ebrei è esattamente parificabile. Credo che gli antisemiti di tutti il mondo brinderanno. Questa svolta del Parlamento italiano è veramente incomprensibile, e lo è a maggiore ragione quando si cambiano le carte in tavola

e vergognosi rispetto a quanto è maturato nella storia dei popoli e di questo Parlamento, per quanto riguarda l'Olocausto,

parlo di eventi che già esistono e sono pronti a creare problemi, riflessioni e discussioni. Certamente, in questo disegno di legge noi andiamo a mettere un un peso su quella che è comunque la discussione, la ricerca, l'esigenza stessa di portare delle prove per quello che si dichiara o che ci si rifiuta di ammettere.

un accertamento dei fatti con una sentenza passata in giudicato, e ad opera di un tribunale internazionale e non di uno qualsiasi. In un qualsiasi Paese dalla sovranità riconosciuta, infatti, si potrebbero celebrare processi con una finalità puramente politica, per ottenere una sentenza che imbavaglia la discussione e impedisce la ricerca. Quindi, io non solo chiedo di sottoscrivere questo emendamento - ringrazio i colleghi che hanno fatto sopravvivere quello che, per me, è non un dettaglio della legge, ma l'unico

Signora Presidente, visto che la precedente richiesta di una spiegazione al parere contrario non ha avuto una risposta, deduco che si è detto di che si è detto di no perché si è concordato questo testo con l'altro ramo del Parlamento, e in particolare con la Presidente della Commissione giustizia che su di esso non ha

almeno a casi che hanno una certa notorietà. In caso contrario, rischiamo di considerare episodi, magari sconosciuti ai più e la cui realtà è ancora da accertare, che rientrano, dal punto di vista della fattispecie (non dal punto di vista della realtà),

bombardamenti fatti senza criterio o addirittura con il criterio di colpire deliberatamente civili non coinvolti nei combattimenti, rischiamo di avere sentenze.

di reati, i quali sono inclusi. Ma almeno si deve stabilire che il reato sia stato accertato da una sentenza di tribunale, per non entrare nella discrezionalità più sfrenata che, innanzitutto, svilisce l'intendimento e, poi, getta nella più totale incertezza sia il giudice che deve essere chiamato a giudicare, sia tutti coloro che intendono fare delle affermazioni di carattere storico, politico, storiografico o anche di propaganda di parte, che è legittima.

un paradosso: se lasciamo il testo così, diamo un potere discrezionale ai giudici che - ahimè - avranno qualche problema a utilizzarlo, tanto che poi qualcuno verrà qui e si lamenterà del fatto che i magistrati applicano le leggi che abbiamo approvato. Se vogliamo evitare questo, dobbiamo arrivare a stabilire delle verità di Stato, esattamente come chiede l'emendamento in base ad esse magari in maniera retrospettiva mandiamo in galera pure Émile Zola, perché con questa legge ci sarebbe andato. Io vi dico fermatevi, perché francamente

e per quelle di libertà, fatte valere poco prima dal collega Quagliariello. Non possiamo perdere l'occasione per segnalare come quel ruolo di accompagnamento alla legislazione, che il Governo avrebbe dovuto svolgere attraverso l'istituto dei pareri e delle motivazioni, sia completamente assente da questo dibattito. E ciò autorizza

perché non avrebbe potuto mettere in moto il processo di revisione. Se vogliamo parlare di vicende ancora più tragiche, tutta la migliore gioventù polacca, tutta l'intellighenzia degli ufficiali polacchi venne sterminata nella foresta di Katyn

sancisce un verdetto, a quel punto lo dobbiamo prendere, nella ricerca storica, come oro colato o, come tutte le cose umane, può essere soggetto a rivisitazione? Ed è ancora peggio

incaricato di tutelare di diritti umani quando c'era ancora Gheddafi. Allora, se uno di tali organismi internazionali dovesse giudicare - ad esempio - Israele sulla base delle considerazioni più volte svolte in questa sede, noi saremmo paralizzati perché nessuno potrebbe più mettere in discussione la sentenza di un magistrato.

Ricordo, ancora una volta, che la verità assoluta sui fatti della storia è propria dei regimi. Sono i regimi - comunisti, nazisti e fascisti - che hanno la verità di Stato. Non esiste una verità di Stato su migliaia e migliaia di casi come quella che voi, in questo caso, avallate anche senza le sentenze dei tribunali nel momento in cui impedite di verificare e approfondire migliaia di fattispecie collegate con i crimini di guerra. Questo è il motivo per cui votiamo contro l'emendamento

quello che stiamo discutendo non è il frutto di mesi di lavoro della Commissione, votato pressoché all'unanimità dal Senato qualche mese fa. Quello che stiamo discutendo è un testo "canguro" presentato nella notte dal Presidente della Commissione quindi, ripercorriamo i fasti del canguro delle unioni civili e del canguro dell'omicidio stradale. In questo caso, per fortuna, non è stata posta la fiducia ma, ancora una volta, il Governo si rimette all'Aula della Commissione in tutto l'*iter* legislativo del provvedimento;

ostilità; - lanciare deliberata mente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti; - il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati

per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari. Colleghi, stiamo parlando di 6 milioni di persone deportate nei campi di sterminio e con

rispetto a chi le ha messe in atto, essendo accusato - come ho dimostrato - di averlo fatto per ragioni etniche o razziali (mi riferisco sempre a Israele). Mi domando ora come si faccia a mettere sullo stesso piano l'Olocausto e queste fattispecie,

ora l'emendamento 1.401 che, se approvato, preclude tutti gli altri emendamenti.

che ha messo in evidenza la verità. Qual è il primo punto da cui occorre partire? Mi permetto di richiamare l'attenzione dei senatori, per lo meno di quelli interessati, perché il dibattito ha registrato interventi di colleghi che hanno parlato senza nemmeno aver letto l'emendamento e il testo che dobbiamo approvare. Il primo punto di partenza concerne l'accusa di una modificazione addirittura integrale del testo

si apprende che l'avverbio «pubblicamente» era stato inserito dal Senato soltanto nell'articolo 1 della cosiddetta legge Mancino-Violante del 1975. L'articolo 1 non fa alcun riferimento al negazionismo, ma si limita a punire soltanto l'istigazione alla discriminazione, ovvero l'istigazione, la propaganda e l'incitamento alla violenza in maniera del tutto generalista. chi ha detto che l'eliminazione dell'avverbio «pubblicamente» avrebbe determinato una dilatazione dell'applicazione del testo che ci interessa (che in realtà è l'articolo 3-*bis*), non ha nemmeno letto il testo su cui l'emendamento incide. L'articolo 3-*bis,* che è l'unico da sempre destinato alla materia del negazionismo

quale attributo dei sostantivi propaganda, incitamento e istigazione. La modifica del mio emendamento è consistita nel sostituire alla la ben più evoluta e costituzionalmente orientata espressione: «in modo da cagionare concreto pericolo di diffusione».

il codice penale sa che la prima risorsa che si può usare in questi casi è utilizzare espressioni proprie della tradizione della giurisprudenza della Corte costituzionale, mentre rispetto al pubblico ci dobbiamo confrontare sulla realtà invece di parlare di cose che non hanno senso - quest'espressione sostituisce alla presunzione di pericolosità di un'espressione pronunciata in pubblico un «concreto pericolo di diffusione». Quindi, vi è un aumento del tasso di garanzia, perché taluno può parlare in pubblico in un contesto nel quale il pericolo di diffusione è escluso, ma tale variante impone che il pericolo sia accertato dal giudice. costituisce un concreto pericolo che il giudice deve accertare. L'espressione utilizzata, ben più evoluta rispetto a quella facilmente immaginabile dell'espressione che si condensa nell'aggettivo «pubblico»,

che ha preceduto la seduta di Assemblea i telegiornali davano notizia di incitamenti a farsi esplodere con cinture imbottite di esplosivo che, utilizzando il *web*, taluno comunicava ad altri. Queste espressioni hanno dato luogo ad un'operazione di polizia giudiziaria che si è giovata proprio dell'assenza dell'aggettivo "pubblico" e dell'avverbio "pubblicamente", che sta nell'articolo 1 della legge Mancino-Violante. Questo per significare che, in un contesto di questo genere, l'eliminazione dell'avverbio "pubblicamente", che era stato inserito dal Senato, risponde ad un'esigenza di tutela della collettività, che è paradossale non sia stata apprezzata in questo dibattito. Noi possiamo avere punito determinate condotte e compiuto attività investigative perché questa legge Mancino-Violante, che è la legge sul terrorismo interno del 1975, eliminando il termine "pubblico", ha consentito di colpire condotte che nessuno può seriamente dire siano compiute in pubblico. Infatti, allorquando taluno incita alla violenza, agli omicidi, alla discriminazione e all'odio razziale attraverso gli strumenti telematici, certamente non lo fa pubblicamente. E allora è un paradosso che il Senato, anzi parte del Senato, sia insensibile a queste esigenze di tutela della nostra società, per tanti versi contraddittoriamente poi a gran voce strombazzate quando queste manifestazioni soltanto esteriori servono a dimostrare che si è in qualche modo interessati a tutelare la sicurezza nazionale. nazionale. Se quello che dico è vero - ed è vero, sol che si legga la pagina del disegno di legge che stiamo approvando, laddove si mettono a confronto il testo del Senato e il testo della Camera - e se questo confronto si arricchisce della lettura del mio emendamento, si capisce che in materia di negazionismo questo testo è soltanto più evoluto, per quell'espressione che ho citato, rispetto al testo licenziato dal Senato, dal quale non differisce in alcun modo. Sono francamente sorpreso e vorrei che qualcheduno mi invitasse ad un convegno nel corso del quale dimostrare il contrario (ci sarebbe davvero da ridere). Questo testo si distingue per aver eliminato quel "pubblicamente" che io mi rendo conto, in un contesto di tranquillità sociale, in un contesto di assenza di pericolo di terrorismo, si potrebbe anche introdurre, ma che, in un momento del genere, sarebbe manifestazione di grave irresponsabilità e di indifferenza assoluta nei confronti degli interessi nazionali pensare di poter eliminare. siccome il testo che proponiamo non differisce in nulla, se non per l'uso di una espressione più evoluta, costituzionalmente orientata, capace di colpire condotte che non saranno mai qualificabili come pubbliche, le critiche mosse a questo testo sono le stesse che si possono muovere al testo da sempre licenziato dal Senato. Chi ha parlato criticando questo testo ha criticato se stesso. È un qualcosa di francamente sorprendente che taluno si alzi per criticare un testo che è in tutto e per tutto identico al proprio, se non più evoluto per la parte che ho detto. È identico anche in quella parte - e qui vado ad una conclusione che accelera un percorso di argomentazione che avrebbe potuto anche essere più lungo, ma che avrebbe stancato, dopo tante cose inutili che sono state dette - in cui si dice che l'incitamento, la propaganda e l'istigazione sono puniti a condizione che essi si fondino sul negazionismo. Questa è una cosa che non si può trascurare di considerare, non soltanto sul versante della sua perfetta identità al testo del Senato. Chiunque ha il testo del disegno di legge può o meno

Insomma, questo testo limita il dibattito scientifico-culturale? No (la risposta è categorica), perché in questo caso non si punisce il negazionismo, ma l'istigazione a delinquere e a commettere gravi delitti

come esemplificazione concreta di ciò che si punisce - «Uccidete il popolo ebraico perché la Shoah se la sono inventata loro». Questa sarebbe condotta riconducibile nel perimetro della punibilità: istigazione a delinquere fondata sulla negazione della Shoah. Ma se non si istiga a delinquere, qualsiasi forma di negazione, di critica storica, politica, culturale, non è minimamente aggredibile da questa disposizione*.

significa che la portata emendativa del testo che noi stiamo votando è assai meno marginale di quello che pare a lui.

già nell'articolo 1 della legge Mancino-Violante, il senatore D'Ascola può benissimo rimproverare a noi

(può darsi), ma, collega D'Ascola, che c'è di male? Questo è il parlamentarismo! In Parlamento si ha il diritto di dissentire, di pensarla diversamente. Non è il mio caso, perché (lo rassicuro), in nome della libertà corporativa della storiografia, in prima lettura anch'io, come il collega Gotor, avevo votato contro questo disegno di legge. Ma il punto è un altro: la ragione è di metodo. Maggioranza e opposizione sono sullo stesso piano; non ci può essere una furbizia consentita alla maggioranza solo perché è maggioranza. Quando abbiamo fatto la discussione generale sul disegno di legge, senza alcun sopracciò da parte del Presidente della Commissione,

allora, inserire un emendamento che ci porta addirittura a non poterci esprimere, come Senato, nel voto finale sul disegno di legge? Non ha senso. Ci sono dei casi nei quali l'opposizione merita rispetto. Il senatore D'Ascola, delle cui argomentazioni ho il massimo rispetto scientifico, accademico, logico, ma non altrettanto parlamentare (perché non ci ha detto che l'emendamento non è stato delegato al Governo, che non è stato delegato al relatore, e che se lo è attribuito lui come Presidente della Commissione), consenta a noi, che non abbiamo mai creduto che il sospetto fosse l'anticamera della verità, di pensare che ciò sia avvenuto perché sul «Corriere della Sera» del giorno prima c'era una sguaiata intervista della Presidente della Commissione giustizia della Camera, che ha avuto anche la trivialità di fare il nome di un collega, il senatore Caliendo, che avrebbe meritato la massima solidarietà sia del Presidente della Commissione sia del Presidente del Senato. E perché il Presidente della Commissione giustizia del Senato di rincorrere l'ennesima mediazione tra Camera e Senato? Del resto, signor Presidente, tutto questo ha avuto conseguenze nei nostri lavori. Io non potrò pronunziare una dichiarazione di voto a nome del nostro Gruppo su questo disegno di legge. Noi ci eravamo espressi in Assemblea, con un intervento del collega Liuzzi, a favore di questo dettato normativo. E io ho troppo stima del collega Liuzzi ed ho troppo disgusto e disprezzo del negazionismo. Il terrorismo non c'entra niente, non facciamo confusione: noi abbiamo combattuto il terrorismo delle Brigate rosse rispettando la libertà di opinione. Se siamo scivolati sul filo - direbbe Malan - del reato di opinione, è proprio perché abbiamo introdotto queste valutazioni improprie, che non avrei voluto ascoltare a proposito di un disegno di legge come questo,

contrario all'emendamento e di astensione sul provvedimento, diventa a questo punto soltanto di astensione, avvalendoci della furbizia

è amaro sentirsi dire il martedì che la richiesta non è pervenuta o che è già stata valutata, quando vi abbiamo ammesso i subemendamenti giovedì mattina alle ore 11. Questo non è un segno di rispetto non dico dell'opposizione, ma dei lavori dell'Assemblea.

e proprio confronto sull'intenzione del Governo e della maggioranza, senza nulla togliere al valore del Presidente della Commissione giustizia e alla correttezza del suo comportamento. Si è voluto inserire un emendamento che diventa sostitutivo dell'intero provvedimento, così vanificando

La modifica era stata disposta e condivisa dalla Commissione giustizia e prevedeva il termine «pubblicamente» in tutti i fatti che rappresentavano e costituivano la condotta di cui all'articolo 3 della legge n. 654

si può discutere veramente sul contenuto del testo, come è stato fatto. Quindi, trovarsi oggi con un provvedimento come quello di cui discutiamo e che siamo chiamati a votare crea anche un imbarazzo e non lo nascondo.

Solo l'evolversi del tempo e un'apertura nuova da parte degli storici che hanno cercato di dire che la ricerca storica non deve essere politica, non deve avere delle influenze o inclinazioni, che possono essere di destra o sinistra o di qualsiasi Noi riteniamo che la storia debba avere la più ampia libertà di studio e purtroppo lo studio della storia può arrivare proprio a discutere sull'esistenza o meno di certi episodi e degli accadimenti. Gli apporti fatti da esimi studiosi in sede di audizioni non fanno che confermarlo. In questi ultimi giorni si parla di altro sui giornali, ma non dimentichiamo il clamore che era sorto attorno a questo provvedimento. È forse troppo facile pensare di votarlo oggi senza creare un grande scompiglio, ma ricordate la discussione che è sorta proprio tra gli storici e gli studiosi che dicevano di fare attenzione a prevedere delle norme come questa. questa. La ricerca storica non può andare in un tribunale. Forse il negazionismo può essere una menzogna e lo è, a volte, ma di certo non può essere un reato in sé.

perché francamente abbiamo assistito a due eccessi. Quella che è andata "in onda" la scorsa settimana è stata presentata come una soluzione di compromesso residuale, di compromesso sul compromesso, e ciò è stato fatto addirittura dai banchi del Governo.

addirittura i pericoli del terrorismo internazionale per giustificare l'emendamento che stiamo votando. Signora Presidente, il compromesso è il più nobile atto in politica, a condizione però che si colga l'oggetto, perché altrimenti rischia di creare pericolose fibrillazioni, come quelle a cui abbiamo assistito, con un riflesso burocratico da una parte l'elevazione dei toni e la dilatazione dell'oggetto stesso dall'altra.

legge - laddove c'è puzza di reato di opinione è infatti bene prendere le distanze - che la norma, oltre ad avere una dimensione penale, ha anche una dimensione è difficile pensare che il senso comune ritenga che la pubblicità o l'incitamento possano avvenire senza o a prescindere dal concreto pericolo di diffusione. È evidente che la dimensione pubblicitaria comporta una necessità di diffusione ed è evidente che questa legge, comunque, indirizza il giudice verso una direzione, che ritengo obbligata. però, signor Presidente, che il problema di fondo sia un altro e cioè che si voglia trovare una soluzione trovare una soluzione nell'ambito penale ad un problema che, invece, è di natura culturale o educativa. Questo è il problema di fondo. Questo è il motivo per il quale questa legge è sbagliata. Questa legge ci porta a mettere nel mirino le opinioni in ogni caso, anche se si tratta di incitamento. Ma perché l'incitamento terroristico contro lo Stato di Israele dovrebbe avere una aggravante se qualcuno lo fa negando la Shoah? Oggettivamente, quello che va punito è il proposito di distruzione dello Stato di Israele così come di ogni altro Stato, indipendentemente dalle ragioni che supportano questo obiettivo criminale. Signora Presidente, proprio perché si vuole dare una soluzione penale a un problema culturale si rischia, dal punto di vista culturale, di compiere una sgrammaticatura che è evidente e che, non a caso, è stata sottolineata da tanti storici. La si può pensare come si vuole, ma la Shoah e l'Olocausto sono una cosa; i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra sono un'altra cosa. Da una parte c'è un fatto accertato

è aperto. È un dibattito non compiuto. Quindi, qui noi ci troviamo di fronte a un bivio. O diciamo che affidiamo a un magistrato il giudizio su determinati fatti, trasformando il giudice in storico; oppure andiamo a ricercare delle verità di Stato che oggettivamente fanno fanno a pugni con i principi propri del liberalismo. Ma il problema è un altro, signora Presidente. Indipendentemente dalle dimensioni, la Shoah viene considerata, dalla cultura diffusa e anche dalla storiografia, un fatto unico e irripetibile. E come si può mettere un fatto unico e irripetibile accanto a fatti vari ed eventuali? Mi consenta un ricordo personale, risalente a una delle ultime discussioni che ebbi con il mio maestro François Furet. Era da poco

di un allievo, che diceva che i crimini del comunismo erano, dal punto di vista numerico, ben maggiori di quelli perpetrati dal nazismo attraverso l'Olocausto,

Stalin avrebbe smesso di perseguitarlo; se invece un ebreo fosse andato in Groenlandia, non sarebbe per questo uscito dall'obiettivo di Hitler. Questa è la differenza che c'è tra la Shoah e quell'elenco di altri crimini e situazioni storiche deplorevoli che il senatore Giovanardi ha elencato. Dunque mettendoli insieme

che è unico e incredibilmente profondo nella sua radice maligna, a tal punto che chi conosce la letteratura sulla Shoah, chi ha letto i libri di Primo Levi e di Semprun, ha trovato addirittura leggeri alcuni capolavori della nostra cinematografia come «La vita è bella» o «Schindler's List», perché non in grado di offrire fino in fondo la profondità di quel dramma storico. Ecco, signor Presidente, questa legge - che non ho votato nemmeno in prima lettura - corre tra le altre cose anche questo rischio. In un colpo solo introduce o sfiora il reato di opinione; concede un incredibile potere discrezionale al magistrato o, in alternativa, spinge verso l'accertamento di verità di Stato; relativizza l'unicità di un fatto storico come la Shoah. Essere riusciti a fare queste tre cose con un semplice disegno di legge e perlopiù da un solo articolo, è certamente un capolavoro per il quale vanno fatti i complimenti alla maggioranza, ma è la ragione per la quale personalmente non voterò questa legge. Signor Presidente, la discussione su questo tema ormai dura da anni e conferma la difficoltà a normare una materia di questo genere per il suo confine incerto e labile, come è la libertà di opinione.

e di un'azione altrettanto forte nell'affermazione dei diritti di libertà e di rispetto dell'umanità da parte di tutti. Non ho quindi cambiato idea rispetto alla mia opinione iniziale, che mi vedeva contrario a una legge su questa materia,

Credo che le prese di posizione pubbliche, anche recenti, di autorevoli storici e intellettuali, anche del mondo ebraico, ci dovrebbero richiamare a una prudenza e a una riflessione ulteriore, perché qui - come dicevano già alcuni colleghi - più che intervenire con il codice penale bisognerebbe intervenire con la formazione dei cittadini nell'accrescimento della propria conoscenza civica e nel rispetto degli altri

ma nello stesso tempo volendo confermare la mia autonomia di giudizio su questioni particolarmente delicate che riguardano la prospettiva non soltanto di questa maggioranza e di questo Parlamento, ma della Nazione. Quest'ultima deve saper distinguere tra principi fondamentali da difendere sempre e azioni legislative che molto spesso mettono in risalto convenienze e opportunità

seguente. Sono quasi dieci anni che il Parlamento discute dell'introduzione di una norma che sanzioni severamente condotte abominevoli quali la negazione di gravissimi crimini contro l'umanità, proseguita per di più con l'intento di istigare all'odio. La prima proposta risale addirittura al 2007 (c'era il governo Prodi) e non se ne fece nulla. fece nulla. A distanza di quasi dieci anni, credo sia arrivato il momento di votare questo provvedimento. Il Movimento 5 Stelle condivide l'opportunità di approvare una norma che possa aiutare a contrastare la preoccupante diffusione di razzismo e di antisemitismo e, in particolare, la negazione di fatti storici ampiamente documentati, quali lo sterminio degli ebrei e di altre minoranze. Noi abbiamo fatto la nostra parte e crediamo sia giunto il momento di concludere l'*iter* del provvedimento in esame. Certo, ci siamo anche assunti

e avevamo ragione. L'intero Senato (cioè sostanzialmente tutti i Gruppi) ci diede ragione rinviando nuovamente il testo in Commissione per essere modificato.

Sarebbe stato un errore enorme. Ricordo che il tutto era stato fatto per celebrare con un voto, auspicato dall'allora presidente della Repubblica Napolitano, la ricorrenza del rastrellamento del ghetto di Roma. Certamente abbiamo avuto ragione nel chiedere allora ulteriore tempo di riflessione, perché il testo inizialmente proposto dalla maggioranza era profondamente sbagliato, come è stato riconosciuto da tutti. Tuttavia non sono pervenute le scuse di chi in quell'occasione per questo motivo ci accusò di xenofobia.

commettendo quindi un doppio errore. Non vi è dubbio alcuno che il più efficace contrasto al drammatico aumento di forme di negazione di fatti storici incontrovertibili come la Shoah

che voglia anche essere un forte richiamo a non dimenticare, oltre che un elemento di dissenso per quelle forme di negazionismo che rappresentano uno degli aspetti più odiosi delle pratiche razziste, fin troppo spesso legate a finalità politiche, in cui la critica della realtà è diretta a procurare e fomentare l'odio razziale. Venendo al provvedimento in esame, non possiamo che fare alcune brevi considerazioni.

luogo,il testo ricevuto *ex novo* in Aula in avvio di seduta avrebbe potuto e dovuto probabilmente essere ben più dibattuto: un'ora per la presentazione dei subemendamenti è tutto ciò che è stato concesso al Parlamento. luogo, il lavoro di accertamento della verità delegato ai giudici con il presente provvedimento, senza nessuna indicazione circa i fatti indicati nelle sentenze pronunciate da organi di giustizia internazionali, rischia di conferire un mandato troppo ampio, quasi a voler scaricare sulla magistratura il mancato coraggio della politica ad adempiere fino in fondo al proprio ruolo. Insomma, se fossimo maggioranza e questa norma l'avessimo proposta noi, l'avremmo formulata come aggravante di reato presupposto e modificata nei termini esposti e, con tutta probabilità, licenziata anche da qualche anno. Siamo tuttavia ben consapevoli di non essere in maggioranza e diamo comunque atto che la proposta presentata dall'emendamento D'Ascola ha l'indiscusso vantaggio di non scalfire l'efficacia della legge Mancino nella sua portata più generale. Consideriamo positivamente anche il fatto che su questo testo ci possa essere un'ampia convergenza politica, auspicata in entrambi i rami del Parlamento, trattandosi di una norma importante, non solo e non tanto per la sua portata normativa, quanto piuttosto per il messaggio chiaro in essa contenuto e che viene, suo tramite, inviato al Paese. Consideriamo inoltre che il testo proposto, che certamente non è il migliore possibile, sia comunque sufficientemente equilibrato e rappresenti dunque, un'efficace via d'uscita ad una *impasse* che dura in Parlamento ormai da troppi anni. Per tutti questi motivi dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Signor Presidente, mi trovo davvero in una situazione in cui speravo di non trovarmi.

ed è a quel voto che mi riferisco per indicare la volontà del mio Gruppo rispetto a questo disegno di legge.

L'unico testo che è legittimato da un voto, il testo sul quale ci dovremmo esprimere, è quello approvato dalla Commissione, all'unanimità per di più. Ebbene, siamo liberi, abbiamo il diritto di esprimerci su quel testo? Abbiamo il diritto di dire che il testo approvato all'unanimità dalla Commissione è quello che preferiamo? Direi di sì, visto che è stato approvato, per l'appunto, dalla Commissione e che in questo momento è in discussione. È stato però presentato l'emendamento del senatore D'Ascola, interamente sostitutivo dell'articolo 1. Sono cose che capitano, a volte anche quando

Io vorrei potermi esprimere contro questo emendamento perché lo riteniamo, come abbiamo ampiamente illustrato anche in sede di votazione dei subemendamenti, fortemente peggiorativo di quanto approvato all'unanimità in Commissione. Vorremmo essere liberi di poterci esprimere su quello che resta e cioè, a questo punto, il testo D'Ascola, dato che sembra abbastanza definito che la maggioranza di Governo approverà questo emendamento. Io vorrei che il mio Gruppo e che ciascuno di noi si potesse esprimere sul testo perché ora la scelta dovrebbe essere tra il testo della Commissione e la proposta D'Ascola. Una volta che la proposta D'Ascola fosse approvata, e verosimilmente lo sarà, dovremmo dovremmo poterci esprime sulla scelta di avere il testo D'Ascola o non avere nessuno testo. In questo secondo caso credo che, probabilmente con dissensi nel nel mio Gruppo, sarei a favore di quel testo: meglio un testo che ha molte carenze che nessun testo. Comunque, al di là di quello che posso pensare io o può pensare il mio Gruppo, deve essere un diritto del Senato potersi esprime su un emendamento essere libero di poter dire che preferisce il testo base, ripeto approvato all'unanimità dalla Commissione, rispetto a quello proposto dall'emendamento D'Ascola, per poi potersi esprimere nella scelta tra il testo così emendato e nessun testo. Di questa procedura, francamente,

di un testo approvato dalla Commissione, quale unico testo del disegno di legge. Se anche fosse, dovrebbe prevalere la possibilità di esprimersi non su un testo qualsiasi succedere che un emendamento sia precluso, ma che sia precluso il testo della Commissione è follia - ma a favore del testo della Commissione. Sono libero di dire, come dico - ed entro ora nel merito - che l'emendamento che stiamo discutendo, e che però costituirà, se approvato, l'intero disegno di legge, ci lascia alquanto insoddisfatti. Veniamo alle differenze principali.

discrezionalità; dunque, meno certezza del diritto: esattamente l'opposto di quanto ci si prefiggeva. In secondo luogo, è stato respinto il sensatissimo emendamento che chiedeva perlomeno di ridurre l'applicazione della norma nel caso dei crimini di guerra - che a mio parere sono troppo numerosi così come inquadrati nell'attuale testo

in questo tempo in cui i pochissimi sopravvissuti a questa mostruosità sono sempre più anziani - e l'inevitabile passare degli anni fa sì che siano sempre meno numerosi che questa memoria non sia soggetta al pericolo di cancellazione. Era opportuno mettere nella nostra legge un sigillo che ponesse rimedio alla mostruosità che si svolse proprio in queste Aule parlamentari, nel 1938, con l'approvazione delle leggi razziali che sono un orrore, una macchia di infamia sul nostro Paese.

Presidente di Commissione, e non mi riferisco al presidente D'Ascola, ma ad altro Presidente di Commissione giustizia di un altro ramo del Parlamento, sommato, è libera di esprimere ciò che vuole. Noi, però, dovremmo essere liberi di procedere nel nostro lavoro, e se abbiamo detto sì all'unanimità ad un testo in Commissione, dovremmo avere la dignità di dire sì allo stesso testo anche in Aula,

di quello della Commissione è che bisognava raggiungere un compromesso di maggioranza tra personalismi emersi in altra parte del Parlamento. Con profondo rincrescimento, annuncio pertanto che il Gruppo Forza Italia non parteciperà a questo voto

Non vogliamo votare contro un testo che diventa obbligatoriamente l'unica cosa su cui ci si può esprimere. C'è un testo della Commissione su cui non ci possiamo esprimere, in quanto dobbiamo esprimerci su un altro

essendo interamente sostitutivo dell'unico articolo del disegno di legge in esame, comporta, con la sua eventuale approvazione, la sostituzione del testo

Infatti, in caso di approvazione del nuovo testo interamente sostitutivo di quello in esame, l'eventuale votazione finale costituirebbe una violazione del principio del *ne bis in idem*, votando due volte sulla stessa cosa. stabilisce, infatti, che quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge,

il cammino è lungo e si collega idealmente a una pagina buia della storia del nostro Paese: mi riferisco alle cosiddette leggi razziali

anni e mesi, delle culture dell'odio e della violenza ci siamo posti il problema di come intervenire e quale strada utilizzare.

contro questa realtà presente oggi in Italia, in Europa e nel mondo, con gli strumenti della cultura, dell'educazione, del confronto democratico, della libera espressione e della capacità di persuasione, che è l'arma fondamentale che esiste in una democrazia. Invece, contro quelle forme di odio che vengono definite in modo molto concreto nella norma che vi viene proposta, propaganda, di istigazione e di incitamento, e che sono orientate a produrre dei delitti (delitti, cari colleghi!), di fronte a questa realtà, come ci viene proposta oggi nella nostra società, allora sì che si può ricorrere all'arma del diritto penale. È la scelta che è stata fatta. E questa scelta, cari colleghi, non è stata fatta con un colpo di mano in Aula, ma è stata fatta raccogliendo l'elaborazione e il lavorìo che abbiamo prodotto proprio qui al Senato, a partire dalla Commissione, e che oggi si racchiude nell'emendamento che ci viene proposto a prima firma del presidente D'Ascola.

Ci sono dei colleghi che adesso criticano questa soluzione; ma si tratta di una soluzione che hanno già votato l'11 febbraio 2015,

Cari colleghi, il testo che abbiamo già votato quasi all'unanimità - e vorrei che tutti i colleghi senatori facessero loro questo esame di coscienza rispetto a quel voto - già conteneva tutte le famose espressioni: «propaganda», «istigazione», «pubblico incitamento»,

Colleghi, questa scelta fu fatta dal Senato l'11 febbraio 2015. Cari colleghi, questa scelta è stata confermata dalla Commissione appena pochi giorni fa; nessun cambiamento è stato apportato su questi punti fondamentali in Commissione; Commissione; ecco perché sembra strano che qui in Aula adesso sorgano dei dubbi su quelle scelte fondamentali che tutti insieme abbiamo fatto, anche con quelli che qui adesso dichiarano il loro voto contrario. Strano. Mi auguro che questo cambiamento sia il prodotto di una legittima convinzione, di una legittima revisione di un'opinione, e non sia invece attirato da uno schematico e - ahimè - povero gioco politico, che spesso non fa onore al lavoro che viene fatto e che viene qui proposto nella sua limpidezza e trasparenza. Dicevo che c'è solo un elemento che viene modificato, l'avverbio «pubblicamente». Cari colleghi, il diritto vivente in questi anni ci ha presentato una realtà che esula dalle categorie del privato e del pubblico. Non volevamo, cari colleghi, entrare nella sfera privata (la famosa cena, che qui più volte è stata rappresentata, dove si esprimono liberamente le opinioni), tantomeno volevamo rinchiudere le scelte che abbiamo fatto dentro la più vasta categoria del pubblico, perché appunto il diritto vivente ci presenta delle fattispecie

quando c'è propaganda, incitamento e istigazione verso i delitti, attraverso una norma molto rigorosa, ben solida, che ci mette in condizione, cari colleghi, di votarla con un'ampia maggioranza, che va al di là della classica maggioranza di Governo. Ecco perché, colleghi, la scelta che abbiamo fatto è molto solida. Il richiamo agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della

se commessi nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili; così i crimini di guerra: quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico su larga scala.

guardino alla propria coscienza e diano conto pubblicamente di questa variazione, sempre legittima, ma - mi auguro - non strumentale ai giochi politici. Scriveremo questa pagina di storia; la vogliamo scrivere insieme e il Senato può andare orgoglioso della votazione che si appresta a fare.

nonostante le mie radicate convinzioni circa la pericolosa ripresa, nella stessa dimensione europea, di sentimenti antisemiti e la necessità di contrastarli in ciascun Paese e con azioni coordinate. La stessa difesa dello Stato di Israele ne è parte essenziale. Ma tutto ciò non può condurmi ad accettare un provvedimento, di cui contesto soprattutto il fatto che esso concorre a un'altrettanto pericolosa estensione della qualificazione penale dei comportamenti umani nel momento in cui dovremmo prendere la strada opposta, secondo criteri di semplicità e di certezza. Riconosco il tentativo di contenimento del danno operato dal presidente D'Ascola, tentando di circoscrivere il campo di applicazione della norma penale. Rimane, tuttavia, ampio il rinvio all'apprezzamento discrezionale del magistrato e soprattutto rimane quel reato di opinione che, per chi ha una qualsivoglia cultura liberale, rappresenta una «contradizion che nol consente».

la questione che vorrei sottoporre riguarda quanto lei ha annunciato e quanto ha annunciato la presidente Fedeli in ordine al fatto che, una volta votato l'emendamento D'Ascola, non si debba procedere ad altra votazione. In realtà, l'articolo 120, comma 2,

che «dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo» - nel caso di un disegno di legge di un solo articolo - «si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge», impone che si voti il disegno di legge.

Adesso siamo in presenza di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 e quest'ultimo, come ha ricordato il senatore Malan, scaturiva da un testo approvato all'unanimità dalla Commissione. Quindi ora, votando l'emendamento, siamo chiamati a scegliere fra due testi nella loro dizione letterale e anche sostanziale. Dopodiché, siamo chiamati a scegliere sul disegno di legge, avendo ascoltato molti interventi, compreso quelli del senatore Quagliariello, se votare a la legge nella sua essenza di introduzione del reato di negazionismo. Una cosa è scegliere un testo (e, come legislatori, dobbiamo scegliere quello che riteniamo più adatto ad essere inserito nel nostro *corpus iuris*); un'altra è fare una valutazione sull'opportunità di inserire una legge di tal fatta nel nostro ordinamento. Quindi mi permetto di invitarla a una riflessione, perché il comma 2 dell'articolo 120, a mio giudizio, indica inequivocabilmente che debba non votarsi l'articolo, in quanto esso è esaurito dalla votazione dell'emendamento interamente sostitutivo; ma lo stesso articolo 120 dice che «si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge». A mio giudizio, dopo aver votato l'emendamento

all'opportunità di non votare un articolo che è già stato così definito, e infatti il «senz'altro» precede il discorso che si voti il disegno di legge, comprese le dichiarazioni di voto. di voto. Adesso, votato l'emendamento, dovremmo votare l'articolo con dichiarazioni di voto: questo sì che sarebbe un doppione rispetto alla votazione finale, perché voteremmo un articolo che è lo stesso del voto finale. Ma dovendo saltare la votazione dell'articolo, come prevede il comma 2 dell'articolo 120, noi abbiamo, signor

ma ritengo di interpretare correttamente il Regolamento con imparzialità. Quando taluni Gruppi hanno fatto una richiesta, a fronte di un importante emendamento del relatore, hanno poi dato atto alla Presidenza di quella seduta della valutazione fatta, ossia di aver consentito ai colleghi di subemendare. Alcuni non sono stati d'accordo, ma mi sembrava una procedura corretta e conforme all'articolo 100 del Regolamento, tant'è che la discussione si è fatta sui subemendamenti, che potevano essere approvati o no, ma questo dipende dall'Assemblea. Adesso, senza

che è già stato approvato. Peraltro, senza scomodare antichi principi di diritto, anche il nostro più moderno Regolamento, all'articolo 97, comma 2, afferma che sono inammissibili gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.

l'Assemblea è sovrana - si proseguirebbe perché l'Assemblea si sarebbe espressa evidentemente immaginando migliore l'altro testo, che non scomparirebbe e sarebbe discusso. La possibilità di far approvare l'altro testo è nelle mani dell'Assemblea, come in tutte le votazioni. La sua richiesta di

che concerne le disposizioni riguardanti la legge europea del 2015 e i due documenti collegati riguardanti le risoluzioni adottate dalla Commissione 14a. Si tratta di un provvedimento urgente perché ci consente di sanare di sanare delle procedure d'infrazione. Credo che, quindi, possa vedersi riconosciuta una priorità rispetto ad altri provvedimenti.

Quindi, secondo me, prima di iniziare la relazione bisognerebbe accertarsi dell'esito della discussione in Commissione bilancio, perché c'è veramente un problema di copertura, tant'è che abbiamo posticipato a domani l'esame completo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la 14a Commissione mi ha dato mandato di riferire a quest'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge europea, così come modificato durante l'esame in Commissione. Ritengo che si tratti di un buon testo, in grado di far compiere un ulteriore passo in avanti al nostro Paese nel rafforzamento della sua posizione in seno al consesso dell'Unione europea. Ricordo, innanzitutto, che l'annuale disegno di legge europea, così come previsto dalle legge n. 234 del 2012 il nostro ordinamento e quello europeo. Un'azione, questa, che avviene attraverso un percorso lungo e elaborato, di cui il disegno di legge costituisce il passaggio finale e formale. Un percorso che passa attraverso molteplici fasi di negoziato gestite dal Governo, in cui il principale interesse di cui si tiene conto è l'interesse nazionale delle nostre imprese, dei nostri cittadini e del nostro tessuto sociale ed economico, seppur nel quadro di un interesse più generale, che è quello dell'Unione europea, che deve essere coesa e funzionale. In questo senso, mi riferisco ad alcuni articoli del provvedimento, che vanno letti a fronte dell'interesse nazionale di riduzione dei casi di contenzioso o precontenzioso con l'Unione europea, senza per questo rappresentare un abbandono della volontà di tutelare e promuovere i diritti, gli interessi e le specificità delle nostre imprese e dei nostri cittadini. Tuttavia, proprio questo secondo aspetto esula dal contenuto proprio della legge europea, così come è stata pensata e architettata

oppure dovrà essere oggetto di azioni politiche da promuovere in sede europea, presso il Consiglio dell'Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione europea. Queste azioni concrete sono intraprese principalmente dal Governo, durante il processo decisionale europeo, ma anche il Parlamento nazionale interviene a pieno titolo, con atti di indirizzo al Governo e attraverso il dialogo politico con le istituzioni europee e lo scrutinio di sussidiarietà sulle proposte legislative che pervengono al Parlamento. Il disegno di legge, presentato al Senato lo scorso 3 febbraio con 22 articoli, si compone ora di un totale di 38 articoli. Di questi, 16 sono diretti a chiudere casi EU Pilot, 4 servono per porre fine ad altrettante procedure di infrazione e 2 a risolvere procedure nell'ambito degli aiuti di Stato. I restanti 16 articoli recano modifiche alla normativa nazionale, al fine di evitare l'apertura di ulteriori casi EU Pilot o procedure di infrazione. Unitamente al disegno di legge, il Governo ha anche consegnato alla Presidenza del Senato, su supporto informatico, gli atti delle procedure di infrazione e dei casi EU Pilot, che sono alla base delle disposizioni di legge contenute nel provvedimento. In relazione a tali atti, il Governo ne ha raccomandato l'utilizzo riservato, in forza del comma 5 dell'articolo 14 della legge n. Secondo gli ultimi dati disponibili, che tengono conto delle decisioni prese dalla Commissione europea il 28 aprile 2016, il numero delle procedure di infrazione a carico del nostro Paese è sceso al minimo storico di 80 procedure, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 18 per mancato recepimento di direttive. Si tratta di un risultato eccezionale, frutto di un lavoro mirato ed efficace, messo in atto dal Governo, con il supporto del Parlamento, che ha portato il numero ad un livello che può essere definito fisiologico, paragonabile a quello degli altri Stati membri. Come è noto, le procedure di infrazione si distinguono in una prima fase (*ex* articolo 258 del TFUE), che si conclude con una sentenza della Corte di giustizia che accerta la violazione e impone la necessaria modifica normativa e il pagamento delle spese giudiziarie. In caso di inadempimento di tale sentenza si può aprire una seconda fase (*ex* articolo 260 del TFUE), che si conclude con un'ulteriore sentenza di condanna, che questa volta comporta il pagamento di sanzioni pecuniarie. Le sanzioni sono di due tipi: la somma forfettaria, che mira a punire l'inadempimento in quanto tale, e la penalità di mora, che ha lo scopo di sollecitare la cessazione dell'infrazione nel più breve tempo possibile. Le due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente nei casi nei quali la violazione del diritto dell'Unione sia particolarmente grave e persistente. Indicativamente, per l'Italia la somma forfettaria minima è pari a euro

Per quanto riguarda la procedura denominata "EU Pilot", essa è stata introdotta sin dall'aprile del 2008, al fine di fornire risposte più rapide e complete a quesiti riguardanti l'applicazione del diritto dell'Unione europea, in particolare quelli rivolti da cittadini o imprese, Il sistema è stato concepito per migliorare la comunicazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri e trovare soluzioni ai problemi riguardanti l'applicazione del diritto dell'Unione europea

che compongono la legge europea, ovviamente in modo sintetico. L'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI relativo alle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. In particolare, con la lettera *a)* si interviene nuovamente sulla disciplina dell'etichettatura dell'olio d'oliva. Con la legge europea 2013-*bis*, sempre nell'ambito del citato caso EU Pilot, si era previsto che «L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo (...), deve essere stampata (...) con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita». Tuttavia la Commissione ha fatto rilevare il contrasto, con la regolamentazione europea, della norma che attribuisce un'evidenza maggiore all'indicazione dell'origine delle miscele degli oli di oliva, rispetto alle altre indicazioni obbligatorie. Pertanto, con la disposizione in questione, si provvede a sanare il contrasto. Con la lettera *b)* si interviene per abrogare la previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. In particolare, la Commissione europea non ha ritenuto conforme alla normativa europea l'indicazione normativa di un termine non superiore a diciotto mesi dell'olio extravergine d'oliva, ritenendo che la qualità di questi oli dipenda da altri fattori e che l'indicazione della durata debba essere lasciata alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità. A quest' ultimo riguardo, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori di oli di oliva, è stato approvato, in Commissione, un emendamento a mia firma, volto a inasprire le sanzioni per l'inadempimento dell'obbligo di indicazione in etichetta della scadenza dell'olio. Sembrano cose noiose, ma in realtà c'è stato un dibattito molto intenso in Commissione. Quindi, credo che siano temi importanti. L'articolo 2 reca una disposizione relativa all'etichettatura del miele, volta a sanare il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato la non conformità, con la direttiva 2001/110/CE sul miele, della norma italiana che prevede, anche per le confezioni importate da altri Stati membri, di mieli raccolti in più Stati membri o Paesi terzi, di indicare obbligatoriamente i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto, senza consentire di indicare solo che si tratta di una miscela di mieli, originari o non originari dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva. L'articolo 3, sull'etichettatura dei prodotti alimentari, è volto a sanare quella parte del caso EU Pilot 5938/13/SNCO relativa alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In particolare, la norma italiana definisce come Paese d'origine «del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e, al contempo, il luogo di origine dell'ingrediente primario. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce, invece, che il Paese d'origine del prodotto è quello definito dal codice doganale comunitario, ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario», che può essere indicato qualora questo differisce dal luogo d'origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione. L'articolo 4 - introdotto durante l'esame in Commissione - reca due novelle di normative di recepimento di direttive europee in materia di dispositivi medici. Le modifiche si limitano a sostituire la locuzione «costi/benefìci» con quella di «rischi/benefìci», a seguito di un'omologa rettifica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 - introdotto durante l'esame in Commissione - estende la sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di sostanze e delle e delle miscele, anche alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, modificativo del precedente. Il capo II del disegno di legge contiene disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.

L'articolo 6 è relativo alle Società organismi di attestazione (SOA). L'articolo 7 riguarda la tassazione delle vincite corrisposte dalle case da gioco.

esclude in ogni caso che l'acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, del personale già impiegato nell'appalto, costituisca trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. L'articolo 9 consente al dipartimento per la giustizia minorile di avvalersi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti competenti, nonché di accedere, tramite tali organi ed enti, alle informazioni contenute nelle banche dati in loro uso.

L'articolo 11 reca norme relative al gratuito patrocinio nei giudizi relativi alle obbligazioni alimentari e nei giudizi relativi alla sottrazione internazionale di minori. L'articolo 12 interviene sulla normativa relativa al permesso di soggiorno per cittadini di Paesi terzi. L'articolo 13 esenta dal pagamento della tassa di circolazione i veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia. L'articolo 14 riguarda il superamento di alcuni profili di incompatibilità tra la normativa italiana e gli accordi comunitari di attuazione dell'accordo di associazione per quanto concerne l'importazione temporanea di autoveicoli. L'articolo 15 L'articolo 15 riguarda l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia. L'articolo 16 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso. L'articolo 17 è volto a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato riguardante le agevolazioni fiscali ai consorzi agrari. L'articolo 18 riguarda la cosiddetta *tonnage tax*. L'articolo 19 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente,

interviene sul trattamento fiscale della raccolta dei tartufi. L'articolo 24 riguarda possibili discriminazioni tra navi di bandiera extracomunitaria e navi di bandiera comunitaria. L'articolo 25 introduce disposizioni sanzionatorie per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie L'articolo 26 reca disposizioni in materia di caccia, finalizzate alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955, in particolare con riguardo alla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. L'articolo 27 interviene sulle disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. L'articolo 28 riguarda il terzo pacchetto energia. Gli articoli da 29 a 34 recano disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. L'articolo 35 intende ovviare a un difetto di coordinamento tra l'articolo 19 e

illustro le risoluzioni presentate e approvate in 14a Commissione su due importanti documenti,

La discussione su questa relazione ha consentito a tutte le Commissioni permanenti del Senato di esaminare i contenuti di rispettiva competenza, non appena il Governo ha provveduto a presentarla Stiamo parlando di uno strumento importante per l'esercizio della funzione di controllo da parte del Parlamento rispetto La prima parte della risoluzione, che riguarda il consuntivo dell'azione del Governo nell'Unione europea, è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali. Si divide a sua volta in tre capitoli: il primo riguarda le due Presidenze del Consiglio dell'Unione europea, della Lettonia e del Lussemburgo, successive a quella italiana; il secondo concerne le questioni istituzionali con particolare riferimento alla cosiddetta *better regulation*, al negoziato sull'ipotesi di Brexit, alla riforma del tribunale dell'Unione europea, alla tutela del *rule of law* dell'Unione Europea, all'adesione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nonché ai rapporti con le istituzioni dell'Unione europea; il terzo capitolo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della crescita economica, delle politiche monetarie, fiscali e di bilancio del piano di investimenti per l'Europa, il cosiddetto piano Juncker, e dell'unione bancaria e dei mercati finanziari.

legiferare meglio e quindi esamina la possibilità di verifiche attente rispetto alle conseguenze e alla gestione delle leggi che l'Unione europea La seconda parte è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali come le politiche per il mercato unico e la competitività, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei capitali e politiche e politiche settoriali, quali le politiche di natura sociale e quelle rivolte al rafforzato di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In questa seconda parte si affrontano nel dettaglio le questioni legate al piano Juncker e ai 315 miliardi per investimenti pubblici La terza parte, rivolta al tema della dimensione esterna dell'Unione europea, illustra le azioni in materia di politica estera il Governo rivendica il ruolo che ha avuto nel 2015, ponendo il Mediterraneo come priorità assoluta della nazione europea e spendendosi per una soluzione politica della crisi libica. Aggiungo che il Governo, sulla cooperazione allo sviluppo, ha insistito nel 2015 sottolineando il nesso stretto tra immigrazione e sviluppo. La quarta parte riguarda l'attività di comunicazione e di formazione relative all'Unione europea e la quinta parte è infine dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee con particolare riguardo al ruolo del comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea e del comitato tecnico di valutazione. Per quanto riguarda, invece, la seconda risoluzione, essa attiene alle priorità dell'Unione europea per il 2016. europea per il 2016. Anche questo lavoro ha consentito a tutte le Commissioni permanenti di esaminare contestualmente tre importanti documenti programmatici annuali: due dell'Unione europea e uno del Governo italiano. Si tratta del programma di lavoro della Commissione per il 2016, che ha un titolo significativo: «È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione»; del programma dei 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea relativo alle Presidenze dei Paesi Bassi, della Slovacchia e di Malta, e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia

da cui è venuto un importante contributo sul merito della risoluzione. Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 conferma strutturalmente la medesima falsariga di quello del 2015, sviluppando e aggiornando le dieci priorità degli orientamenti politici formulati dal presidente Juncker all'avvio della nuova Commissione. Anche l'idea di fondo del programma, che lo scorso anno era espressa con il titolo «Un nuovo inizio», è mantenuta e ulteriormente rafforzata con l'affermazione che è il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. La Commissione, quindi, intende continuare a mettere in atto e guidare un'azione energica, in discontinuità politica rispetto al passato, per fare fronte alle sfide epocali connesse con la crisi economica*,* finanziaria, istituzionale e sociale, aggravata ulteriormente dalla minaccia globale del terrorismo di matrice islamista e da una pressione migratoria senza precedenti sulle frontiere meridionali dell'Unione. Serve cambiare

mia né della nostra Commissione quella di verificare come per tanti cittadini europei l'Europa oggi anziché un'opportunità venga letta come un problema. Vado a elencare le dieci priorità politiche, che poi producono 23 proposte legislative: occupazione, crescita e investimenti, il mercato unico digitale, la costruzione di un'unione sull'energia, il rafforzamento del mercato interno dell'Unione e la base industriale dell'Unione, sostenendo le piccole e medie imprese, l'unione monetaria più equa, l'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, lo spazio di giustizia e diritti fondamentalmente basati su reciproca fiducia, verso una nuova politica dell'immigrazione; un ruolo più incisivo a livello mondiale della politica estera e di sicurezza comune e infine il cambiamento democratico del legiferare meglio, ovvero la questione che ponevo prima: la necessità di mettere in campo verifiche sull'impatto della legislazione europea più cogenti e attente. Queste sono le priorità. Concludo sottolineando il fatto che in entrambi i documenti è evidente che il futuro dell'Europa si gioca su tre questioni fondamentali: come l'Europa saprà

con unità il tema della lotta al terrorismo; in che modo l'Unione europea saprà affrontare il tema dell'immigrazione senza perdere i propri principi e valori. Signor Presidente, ciò che ci ha riferito la senatrice Comaroli corrisponde assolutamente al vero.